poiche´ la Camera dei deputati ha approvato senza modifiche il decreto-legge n. 43, in materia di emergenze ambientali e altre misure urgenti, previsto dal calendario dei lavori, l’Assemblea tornera` a riunirsi domani mattina, alle ore 9,30, per il seguito della discussione di mozioni sul corridoio ferroviario Adriatico, nonche´ domani pomeriggio, alle ore 16, per le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2013. Comunico che sono pervenute alla Presidenza mozioni, interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna. Ordine del